decreti-legge». In data 13 agosto 2011, e` stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze: «Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» Il provvedimento estato deferito alla 1ª Commissione permanente per i presupposti di costituzionalita di cui all’articolo 78, comma 3, del Regolamento

Le predette Commissioni sono fin d’ora autorizzate a convocarsi affinche´ la 5ª Commissione permanente riferisca all’Assemblea a partire dal 5 settembre. La definizione ulteriore dell’iter del provvedimento sara` stabilita da una Conferenza dei Capigruppo da convocare nel corso della prossima settimana.